Onorevoli colleghi, venerdì scorso, si è spenta a Roma, all'età di 87 anni, Susanna Agnelli. Nata a Torino nel 1922, terza figlia di Edoardo e nipote del senatore Giovanni Agnelli fondatore della principale azienda automobilistica italiana, seppe mettere al servizio del Paese le sue straordinarie qualità umane e politiche, le sue conoscenze e il suo grande patrimonio culturale. La sua esperienza e l'impegno diretto al servizio della collettività iniziò con l'elezione a Sindaco del Comune di Monte Argentario nel 1974. Nell'esercizio di quella carica, mantenuta per 10 anni, Susanna Agnelli si distinse per le vigorose battaglie a tutela del territorio e l'efficace contrasto all'abusivismo edilizio. L'anno successivo vide la luce la sua autobiografia nella quale, con il taglio sapiente e raffinato di una scrittrice di talento, condivideva con i lettori i ricordi dell'infanzia torinese, le relazioni familiari e i contatti con alcune tra le figure più significative dell'Italia di quegli anni. Un'opera di valore letterario e storico e, allo stesso tempo, una lezione di stile ed eleganza narrativa che conquistò immediatamente i favori del pubblico, meritando il Premio Bancarella nel 1975. Nel 1976, su proposta di Ugo La Malfa, fu candidata alla Camera nelle liste del Partito Repubblicano, conseguendo l'elezione a deputato per la VII legislatura. In occasione della prima elezione diretta, nel 1979, venne chiamata tra i rappresentanti italiani al Parlamento europeo, dove partecipò ai lavori della Commissione per le relazioni economiche esterne. Al principio della IX legislatura, nel 1983, nuovamente candidata nelle liste del Partito Repubblicano, entrò a far parte della nostra Assemblea e fu quindi chiamata a ricoprire il delicato incarico di Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, che conserverà fino al 1991, in ben cinque compagini governative, dal I Governo Craxi al VI Governo Andreotti. Le qualità dimostrate in occasione di quella lunga esperienza di Governo si riveleranno decisive nel 1995 quando a Susanna Agnelli, prima ed unica donna della storia d'Italia a ricoprire questo ruolo, fu affidato l'incarico di Ministro degli affari esteri in occasione della formazione del Governo Dini. In quella veste si trovò a fronteggiare un difficile quadro internazionale segnato da gravi instabilità regionali, prodotte da crisi sanguinose come quella che scuoteva la ex Jugoslavia e dalla repentina ridefinizione degli equilibri globali dopo la dissoluzione del blocco sovietico, che rischiava di determinare processi rapidi ed unilaterali di riforma del sistema delle Nazioni Unite che avrebbero seriamente compromesso la posizione internazionale del nostro Paese. Il Ministero degli affari esteri guidato da Susanna Agnelli fu allora il principale snodo di uno sforzo di un intero Paese che, proseguito nell'azione dei Governi successivi, anche di segno diverso, ha saputo evitare che si giungesse ad una riforma delle Nazioni Unite e del Consiglio di Sicurezza ingiustamente penalizzante per il ruolo internazionale dell'Italia e in contraddizione con quello crescente dell'Unione europea e di altre realtà internazionali. Alle sue straordinarie capacità organizzative e di persuasione si deve ancora, nel 1990, la costituzione della Fondazione Telethon che, a partire dal dicembre di quell'anno, si occupa di raccogliere fondi per destinarli, attraverso un rigoroso e trasparente meccanismo di selezione della validità scientifica dei progetti, alla ricerca e alla sperimentazione per la cura della distrofia muscolare e delle altre malattie genetiche. Parte essenziale dell'attività della Fondazione, secondo un'intuizione personale di Susanna Agnelli, è orientata a favorire e sostenere il rientro in Italia di studiosi e ricercatori emigrati all'estero per impiantare nel nostro Paese centri di eccellenza per la sperimentazione di nuove terapie. In questi tre ambiti dell'agire umano - la politica, la letteratura, l'impegno sociale - Susanna Agnelli ha desiderato fortemente impegnarsi in prima persona, mettendo il proprio volto, le proprie energie e le proprie capacità al servizio della crescita e del benessere del nostro Paese. Con il suo impegno e con il suo prezioso contributo si è rivelata una delle figure femminili più forti e significative del secolo scorso. A nome di tutta l'Assemblea e mio personale esprimo quindi il più sentito cordoglio e una viva partecipazione al dolore della sua famiglia in particolare alla figlia Samaritana, presente oggi in tribuna con il consorte - e profonda vicinanza a tutti i ricercatori e i dirigenti della Fondazione Telethon, chiamati a perpetuare, nella loro quotidiana azione, la tenacia e la passione del loro compianto Presidente. Invito pertanto tutti i colleghi ad osservare un minuto di raccoglimento.

Susanna Agnelli, nonostante provenisse da una famiglia così importante per il nostro Paese, era una donna semplice, vicina ai problemi della gente. Una donna che si impegnò profondamente nel sociale, cercando con la sua Fondazione di raccogliere fondi per la ricerca. Una donna colta e semplice, la cui attività in favore dei più bisognosi inizia da giovanissima, durante la seconda guerra mondiale, con la Croce Rossa. Il suo era un impegno forte e costante che andava al di là di ciò che potesse rappresentare. Fu una vita, la sua, totalmente impegnata, sia dal punto di vista sociale che politico: sindaco, deputata, senatrice, Sottosegretaria e Ministro degli affari esteri, prima ed unica donna nella storia italiana al vertice In quel ruolo iniziò la battaglia in seno alle Nazioni Unite per impedire che la riforma del Consiglio di Sicurezza potesse portare di fatto all'esclusione dell'Italia dal consesso dei grandi del mondo. Parlamentare europea nel 1979 per le liste del PRI, membro della Commissione per le relazioni economiche esterne, aderì al Gruppo parlamentare liberaldemocratico, rimanendo in carica fino all'ottobre 1981. In quegli anni è stata l'unico membro italiano della Commissione mondiale per l'ambiente e lo sviluppo. La carriera politica di Susanna Agnelli non prevaricò mai la sua attività di scrittrice e di giornalista: una scrittrice e una giornalista dalla prosa semplice ed efficace, perché semplicità ed efficacia erano le doti che la contraddistinguevano e che ce la fanno ricordare con grande stima e affetto. Una donna risoluta e sempre animata dalla voglia di fare bene. Questa era Susanna Agnelli. A lei oggi va il nostro più sentito ricordo. facoltà. LANNUTTI *(IdV)*. Signor Presidente, colleghi, con Susanna Agnelli, sorella prediletta dell'avvocato Giovanni Agnelli, scompare un pezzo della storia italiana. Sindaco, parlamentare, sottosegretario, ministro, Susanna Agnelli dal 1992 era presidente del Comitato Telethon, l'ente che raccoglie fondi per finanziare i migliori progetti di ricerca sulle malattie genetiche rare. Non ha mai tralasciato il suo impegno sul fronte umanitario, che risaliva però all'età giovanile quando, durante la seconda guerra mondiale, entrò nella Croce Rossa per portare il suo aiuto sulle navi che trasportavano soldati feriti. È stata la prima donna italiana a ricoprire l'incarico di Ministro degli affari esteri. Per 10 anni ha ricoperto la carica di sindaco del Comune di Monte Argentario, dove si è impegnata assiduamente nella salvaguardia di quell'angolo di meraviglia naturalistica, che oggi il cemento e l'asfalto stanno fin troppo mortificando. Nel 1976 è stata eletta deputato e nel 1983 senatore nelle liste del Partito Repubblicano. Come Sottosegretario ha fatto parte dei Governi Craxi, Goria, De Mita e Andreotti. È stata membro ONU nella Commissione internazionale per i diritti umanitari e nella Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo. Nel 1984 ha ricevuto la laurea *honoris causa* in legge dalla Mount Holyoke University del Massachusetts e nel 1996 è stata nominata cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana. Sapeva usare le parole, ne conosceva la potenza e lo ha dimostrato con i suoi libri. Il suo racconto della vita di casa Agnelli, "Vestivamo alla marinara" (blu d'inverno, bianco e blu a mezza stagione, bianco in estate), rappresenta un'immagine fedele della borghesia italiana a cavallo tra le due guerre nella cronaca di una famiglia che ha contato molto in Italia: ricchezza e forza industriale; FIAT, cattedrale del capitalismo ed insieme pasto per una marea di dipendenti diretti e indiretti degli stabilimenti e della miriade di attività satelliti della produzione. Donna tenace, che non ha mai vissuto all'ombra della sua famiglia, ha sempre dato tutta se stessa all'impegno umanitario, come la sua dedizione alla Fondazione Il Faro, nata nel 1997 per insegnare un mestiere ai giovani in difficoltà, italiani e stranieri, consentendo loro di acquisire capacità professionali spendibili sul mercato. Non amava andare in televisione, ma lo faceva per dare voce alla ricerca.

E sono ancora meno quelli che lo mettono in pratica». Continuava dicendo: «Quando ripenso a quelle mamme, quando leggo l'impegno e la speranza negli occhi dei nostri giovani ricercatori e quando rifletto sul fatto che tutto questo è stato reso possibile dalla generosità e dalla fiducia di milioni di persone, allora penso che non tutto è perduto e che, a proposito di meritocrazia, forse noi italiani ci meritiamo un Paese migliore». Susanna Agnelli avrebbe potuto occuparsi di qualunque altra cosa: aveva solo l'imbarazzo della scelta. Invece, ha deciso di mettersi a disposizione delle nuove frontiere della medicina e, in particolare, della lotta alle malattie rare.

Con Susanna Agnelli se ne va una donna intelligente, con la sua schiettezza, cui teneva tantissimo, e che le ha procurato spesso fama di donna difficile. A lei va un pensiero rispettoso per tutte le cose buone che ha fatto soprattutto perché, come ogni grande donna, non si è mai risparmiata. Signor Presidente, le commemorazioni, per definizione, mettono in risalto e danno lustro alle virtù e ai meriti di chi è scomparso, lasciando in disparte aspetti discutibili. Chi approda al ricordo del Parlamento, di sicuro ha segnato qualche pagina della storia del nostro Paese. Ebbene, oggi diamo il nostro commosso saluto a Susanna Agnelli, l'ultima conosciuta espressione della storica famiglia e, soprattutto, figura che è entrata nel cuore degli italiani. Mi riferisco alla sua lunga attività alla guida di Telethon, una vera macchina per raccogliere fondi per la ricerca, che ha avuto nella signora Agnelli insieme il faro e l'anima. Questa testimonianza le ha assicurato generale riconoscenza e, soprattutto, ha trasformato un personaggio della più alta borghesia del Paese in una persona amica, vicina a tutti noi. noi. In questi giorni abbiamo letto la sua ricchissima biografia, che va dall'impegno politico e amministrativo

sociale. E' ricordata la sua attività di giornalista e di scrittrice e il suo spazio sul rotocalco "Oggi", quando rispondeva con ironia, saggezza e classe ai quesiti dei lettori. Ma ricordandola come presidente di Telethon mettiamo insieme due aspetti fondamentali e peculiari della nostra gente: il volontariato e la generosità, fondata sul sentimento, sull'attenzione, sull'amore per il prossimo e sull'impegno e l'intelligenza che si fondano invece sulla scienza, sullo studio, ma con l'uguale obiettivo di far del bene all'umanità. Proprio qualche settimana fa festeggiato i 100 anni di un'altra donna, anch'essa piemontese, che della ricerca ha fatto una ragione di vita. Versanti diversi, ma comune spessore in Rita Levi-Montalcini e Susanna Agnelli, che non a caso hanno onorato, e la prima onora tuttora, questo ramo del Parlamento. L'addio di oggi assume perciò il valore profondo della riconoscenza verso chi, avendo avuto natali fortunati, ha saputo farne tesoro, sapendo unire e distinguere insieme la ricchezza materiale e la ricchezza dell'animo.

è stata senatore della Repubblica, ma noi oggi le faremmo un torto se la ricordassimo in quest'Aula del Senato soltanto per quella sua esperienza, sia pure molto rilevante. La sua vita è stata, sino alla fine, così ricca di interessi e di impegni che noi possiamo dire, già da oggi, che Suni Agnelli verrà ricordata come una delle grandi donne del suo tempo, un'autentica protagonista del XX secolo italiano. Crocerossina in Africa durante la Seconda guerra mondiale. Sindaco tenace e coraggioso. Parlamentare. Sottosegretario e Ministro. Azionista rilevante e influente della FIAT. Scrittrice di successo. Un'esistenza tutta segnata da un profondissimo impegno civile e sociale che non delegava mai, ma che voleva e sapeva svolgere in prima persona, sul campo, con iniziative concrete, operative. Questa è stata, nella sua vita, Susanna Agnelli. Una vita lunga, scandita da mille attività, da impegni molto diversi tra loro, tenuti insieme da una personalità molto forte e dallo speciale carattere con il quale ha sempre onorato le responsabilità che le venivano assegnate o che lei stessa si assumeva. Chi l'ha conosciuta sa che in tutto quel che ha fatto Suni Agnelli ha messo l'anima, ha dedicato cultura e sensibilità, energie ed esperienza. Da buona piemontese aveva fortissimo il senso della sua responsabilità civile, dei suoi doveri verso il Paese. Da Sindaco ha difeso - come ha già ricordato

Se tutti i Comuni d'Italia fossero stati amministrati con lo stesso intelligente rigore, con lo stesso rispetto per l'ambiente, con eguale responsabilità sociale, oggi il nostro Paese sarebbe migliore. Da Sottosegretario e Ministro degli affari ha esercitato con straordinaria sensibilità politica, in anni difficili, il complesso mestiere di capo della diplomazia italiana. Lo ha fatto con competenza e, soprattutto, con quella lealtà e quel rigore intellettuale che nelle relazioni internazionali determinano, più di ogni altra qualità, il prestigio e la credibilità delle Nazioni e dei loro governanti. È stata un Ministro affidabile, non solo per i Paesi alleati, ma anche per tutti gli altri Paesi con i quali l'Italia intrattiene rapporti. È stata prima deputato e poi senatore del Partito Repubblicano: fu personalmente Ugo La Malfa a chiederle l'impegno politico. Repubblicana, è stata espressione di un partito al quale la piccola dimensione non ha mai impedito di essere politicamente autorevole, un partito che ha rappresentato in Parlamento un'Italia seria, anche se molto minoritaria. Ricordare Susanna Agnelli, Ugo La Malfa, Giovanni Spadolini e Bruno Visentini, ci spinge ad interrogarci su quanto giovi all'Italia avere oggi leggi elettorali sempre più ipermaggioritarie. Per evitare i danni dovuti all'eccesso di frammentazione, vengono eliminati dalla vita politica pezzi importanti del pensiero del Paese. Non si può parlare di Susanna Agnelli senza ricordare quanto sia stato rilevante nella sua vita l'impegno sociale nella lotta al dolore e alla povertà. Presidente di Telethon, spese la sua autorevolezza nel reperimento delle risorse necessarie a sostenere la ricerca e mise tutto il rigore di cui era capace per impedire la dispersione e lo spreco dei fondi disponibili per la lotta a gravi malattie. Impose, conseguentemente, che le risorse venissero investite esclusivamente sulla base del valore scientifico dei progetti da finanziare. Oggi, dopo decenni, l'Italia comincia ad imparare questa lezione. Amava i giovani, stava volentieri con loro e li ascoltava con attenzione. Nel novembre del 2001 si rivolse al presidente Ciampi chiedendogli aiuto e gli disse: «Signor Presidente, non cacciamo i giovani immigrati. Conosco questi ragazzi e le loro aspettative, spero che lei possa fare qualcosa». Parlava forte della sua esperienza personale. Con la sua Fondazione Il Faro assisteva 130 albanesi, kosovari, iracheni, marocchini, tunisini, romeni, ucraini, che erano arrivati in Italia quando avevano a 15-16 anni con mezzi di fortuna. Aiutava quei ragazzi non solo col necessario contributo economico, ma pretendendo da ciascuno di loro un impegno serio nella formazione professionale, quale unica strada in grado di condurli ad un futuro migliore. Ora che Suni Agnelli è scomparsa, dobbiamo augurarci che il suo patrimonio di generosità trovi il modo e le persone necessari per andare avanti e crescere ancora. Suni Agnelli era una donna molto vitale, curiosa, anticonformista, di grande intuito: tutte virtù femminili. Veniva da una grande famiglia e, a sua volta, aveva voluto una sua grande famiglia, sei figli, a testimonianza di come gli impegni, le responsabilità, la complessità della sua vita non abbiano mai soffocato la sua natura femminile, il suo essere pienamente e profondamente donna. Una volta disse che «senza pazienza non si sopravvive»: parlava certamente di quella pazienza forte, di quella tenacia che è propria delle donne e che noi uomini conosciamo meno. In questi giorni - e mi avvio alla conclusione, signor Presidente - qualcuno dei suoi amici ha ricordato che a Suni Agnelli poteva capitare di essere molto diretta, quasi rude. È vero, poteva essere così, ma non accadeva mai per capriccio. Diventava brusca quando entravano in ballo questioni cui attribuiva grande valore, questioni di principio, morali o civili. Lasciatemi dire che anche questo era un tratto forte della sua femminilità. Sono le donne, più che gli uomini, che spesso con l'esempio ci insegnano a non cedere al compromesso quando sono in gioco le grandi questioni; sono le donne che più frequentemente ci fanno comprendere la necessità di essere intransigenti sui principi. Suni Agnelli ci ha lasciato questo insegnamento. Signor Presidente, colleghe e colleghi, con Susanna Agnelli scompare una donna che ha saputo, nell'ultimo quarto del secolo scorso, interpretare in modo pieno il proprio ruolo di esponente di una grande famiglia di imprenditori e politici, profondamente legata alle vicende italiane. Di lei voglio ricordare l'impegno come amministratore locale, nel ruolo di Sindaco di Monte Argentario, località che ha profondamente amato e per la quale ha speso il proprio impegno pubblico per un decennio, contribuendo alla salvaguardia e alla valorizzazione dell'ambiente naturale, anche anticipando sensibilità e iniziative che a quel tempo apparivano pionieristiche. Una figura decisamente all'avanguardia rispetto all'epoca in cui ha svolto il proprio operato in campo politico e sociale. Ecco perché ritengo debba essere considerata da tutti, in particolare dalle nuove generazioni, un modello da seguire. Un esempio per chi si vuole affacciare al mondo della politica, interpretandola come una missione al servizio della collettività: la politica nel significato più nobile del termine. L'impegno politico di Susanna Agnelli è proseguito nel ruolo di deputato prima, e di senatore poi, tra le fila dei Partito Repubblicano, per approdare infine al Governo come Sottosegretario e Ministro degli affari esteri, unica donna che in Italia abbia mai ricoperto tale prestigioso incarico. Anche sotto questo aspetto, la sua figura ha anticipato i tempi, dimostrando la valenza che le donne possono avere nell'impegno politico, fino ai massimi livelli istituzionali. Nella sua attività alla Farnesina la senatrice Agnelli è stata espressione dell'imprenditoria italiana nel mondo, accompagnando e favorendo l'affermazione del *made in Italy* sui mercati internazionali. Era ella stessa, con la storia personale e quella della propria famiglia, di cui portava il nome con orgoglio, il miglior promotore della capacità d'intrapresa, del dinamismo e dell'inventiva che hanno permesso al nostro Paese di diventare sinonimo di stile ed eleganza in molti settori produttivi: un esempio delle grandi potenzialità di cui l'Italia dispone nell'ambito della creatività nei settori più disparati, nella progettualità anche nella sfera della politica. Conclusi gli impegni istituzionali, la senatrice Agnelli non cessava comunque di ricoprire un rilevante ruolo pubblico, impegnandosi con convinzione nel campo della solidarietà e nella lotta alle malattie genetiche, organizzando in Italia la maratona Telethon che di anno in anno ha riscosso sempre più adesioni, anche grazie ai suoi sforzi, alla tenacia e determinazione che sapeva mettere in ogni attività. Un segno questo del suo impegno sociale che dimostra come la tenacia e il coraggio, tipici di una donna appartenente ad una delle più importanti dinastie imprenditoriali italiane, non fossero disgiunti, anzi andassero di pari passo con una notevole umanità e capacità di dedicarsi agli altri, a chi ha più bisogno. È stato notato che la scomparsa di Susanna Agnelli coincida con un momento particolare per la vita dell'azienda cui la famiglia Agnelli ha legato da oltre un secolo il proprio nome, la più grande azienda italiana, la FIAT, a cui proprio il nonno, il senatore Giovanni Agnelli, volle dare una forte proiezione internazionale. In queste settimane il dinamismo della FIAT fa da contrasto alle difficoltà e alla grave crisi che ha colpito i colossi dell'auto americana, segnatamente *Chrysler* e *General Motors*, tanto da far sperare che l'iniziativa, ancora in corso, dell'amministratore delegato Sergio Marchionne, supportato dall'azionista storico, possa concludersi con la creazione di un polo automobilistico tra i più forti al mondo: un nuovo modello aziendale di ampio respiro internazionale ma che con gli assetti produttivi e decisionali, con i livelli occupazionali - insomma, con la «testa» - resti a Torino. Siamo certi che questo risultato sarebbe stato per Susanna Agnelli il più gradito omaggio e riconoscimento per una lunga vita pubblica, spesa nell'impegno sociale su più fronti, sempre facendosi interprete di quello stile, di quella signorilità, di quel coraggio che in questi giorni di lutto sono stati raccontati e ricordati da molti commentatori come un segnale del tratto così tipicamente torinese, orgoglioso e riservato, cortese ma fermo, che ha contraddistinto la terza generazione degli Agnelli, a partire dai fratelli Gianni e Umberto, entrambi senatori. Ci uniamo al cordoglio dei figli e di tutta la famiglia, profondamente commossi per la sua scomparsa.

per richiamare la notizia che abbiamo appreso da qualche ora in merito alla decisione dei giudici della 10a sezione penale del tribunale di Milano che hanno condannato l'avvocato Mills.

dalle società *offshore,* al fine di eludere il fisco e la normativa anticoncentrazione, consentendo in tal modo anche il mantenimento della proprietà di ingenti profitti illecitamente conseguiti all'estero. Devo manifestare, signor Presidente, un grande disagio istituzionale ed anche politico nel chiedere la parola su questo argomento

all'immunità che ha acquisito con il cosiddetto lodo Alfano. Vede, signor Presidente, la decisione del tribunale di Milano di Milano fa legittimamente sospettare che proprio a questo servisse il lodo Alfano. Credo che il Presidente del Consiglio avrebbe tutto da guadagnare sul piano del prestigio personale e della considerazione internazionale se rinunciasse ad un'immunità che non fa male soltanto a lui ma fa male al nostro Paese. Dal punto di vista politico e parlamentare, pur

l'attuazione di tale decisione credo leverebbe ogni significato parlamentare e politico al gesto che il presidente Berlusconi ha voluto compiere. Le chiedo quindi, anche a nome dei senatori

anche alle considerazioni sviluppate dal senatore Zanda. Anche il mio Gruppo avverte l'imbarazzo nel prendere la parola su una questione che ha un grande rilievo giudiziario, ma anche politico;

dichiarato ad un'emittente televisiva di voler riferire in Parlamento su questa vicenda ciò significa che egli stesso assegna ad essa una

Ciò che non condividiamo

lo ricordo - ha impegnato questo ramo del Parlamento e la Camera dei deputati in lunghe discussioni sul cosiddetto lodo Alfano, cioè la normativa che, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione, ha assicurato la cosiddetta improcessabilità e, di fatto, l'impunità per le alte cariche dello Stato. Stato. Noi riteniamo che quello strappo costituzionale non sia sanabile venendo a parlare in Parlamento di una vicenda giudiziaria; riteniamo che l'unico luogo

valore politico ad una vicenda che è gravemente lesiva dell'immagine del Parlamento e della stessa sua rappresentanza governativa. Ci saremmo aspettati altri gesti, anche più forti, sia pure poi respinti dall'Aula del Parlamento, sia pure poi respinti dal Capo dello Stato: un atto di dimissioni come segnale di valenza politica e non la scelta di un'aula anziché di un'altra. Si fugge da un'aula di giustizia e si dice di voler parlare in una Aula parlamentare. Anche questa scelta riteniamo sia assolutamente impropria e non condivisibile. Comunque, aspetteremo le comunicazioni che il Presidente del Consiglio ma non rinunziamo alla speranza di un sussulto di dignità per cui egli rinunzi al lodo Alfano e vada in un'aula di giustizia a giustificarsi e a difendersi. non saremo certo noi oggi a difendere il presidente Berlusconi, anche perché

e che delegittimi l'attività della magistratura. Se poi queste sentenze provengono da un giudice che, pubblicamente, più volte, si è schierato contro l'attività di questo Governo, è chiaro che i cittadini, gli stessi elettori non possono che avere una visione distorta dell'operato della magistratura; sicuramente ne viene delegittimata l'attività.

questo vogliamo rinnovare una solidarietà politica convinta al presidente Berlusconi. Non voglio entrare in questa sede nel merito di vicende che discuteremo, rinnovando forse la lettura di alcuni articoli e scritti di chi ha giudicato oggi oggi questa vicenda giudiziaria e nel passato - mi riferisco al giudice Gandus - ha scritto pagine che ricordiamo per il carico di spirito di parte che esprimevano. Non abbiamo nessun timore ad un pubblico confronto in un'offensiva di verità

C'è chi fa la campagna elettorale con i comizi, c'è chi la fa pubblicando con una certa tempistica le sentenze. Noi andremo avanti per la nostra strada, convinti che gli ulteriori gradi di giudizio, dove forse ci saranno giudici meno prevenuti, daranno la giusta soddisfazione a chi la merita, e convinti che il giudizio degli elettori sarà in sintonia con quello che in questi anni è stato espresso con convinzione e con chiarezza.

Signor Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo,

è conclusa. Il tempo di solito fa dimenticare, ma quando la vita ti mette di fronte ad eventi dolorosi, come quelli che abbiamo appena vissuto, non si può nascondere la testa sotto la sabbia

non si ripetano più gli errori commessi, perché la gente d'Abruzzo possa tornare a vivere al più presto e perché la terra d'Abruzzo, L'Aquila, hanno diritto di tornare alla vita al più presto.

Prima di affrontare il merito del contenuto del disegno di legge, che tratta la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto in terra d'Abruzzo, vorrei dare atto al Governo, e in primo luogo al presidente Berlusconi, dell'attenzione con cui ha costantemente seguito le vicende delle popolazioni terremotate e dell'interesse mediatico che ha richiamato continuamente su di queste e sull'evento. Vorrei contemporaneamente ringraziare tutti gli operatori del soccorso, che in pochi giorni sono venuti incontro ai dolori e alla sofferenza di quelle popolazioni, mentre da noi ci sono voluti anni. all'Umbria, a quella parte dell'Umbria - come ho detto - che fu particolarmente colpita dal movimento tellurico del 1997 e che, per certi versi, somiglia a quello d'Abruzzo. Posso dire che una delle cose che più temevano coloro che avevano perso i propri cari, le proprie case e quanto possedevano, tra cui il lavoro, era di essere dimenticati.

La ricostruzione divenne fin dall'inizio una parte del bilancio della Regione Umbria, poiché commissario straordinario venne nominata la sua Presidente, valutata solo per la sua capacità di stimolare il PIL (con la ricostruzione doveva crescere il PIL dell'Umbria) e soprattutto di produrre consenso elettorale, grazie a leggi e leggine regionali piene di lacci e lacciuoli e di apertura e chiusura di termini, che significa poi posti in graduatoria alla bisogna. L'ho detto per dieci anni, quindi se qualcuno ha da dire qualcosa sono pronta a rispondere. Voglio far presente ai colleghi del Partito Democratico che osannano quanto fu fatto in Umbria

costantemente Comuni virtuosi, che riuscivano a realizzare progetti ma che dovevano attendere le graduatorie prima di attuarli (ci sono alcuni umbri qui, che lo sanno). La ricostruzione è andata avanti così, a singhiozzo. Il lavoro è stato in gran parte appaltato a ditte provenienti da fuori Regione, si sono riscontrate infiltrazioni mafiose e camorriste, tanto da finire sui giornali anche per questi fatti.

la sensibilità del Governo. Da ciò deriva che gran parte delle aree terremotate risultano desertificate e prive della presenza dell'uomo per la mancanza di occasioni di lavoro e l'assenza di prospettive economiche. I giovani vanno a lavorare nei centri più grandi, con la conseguenza che si sono smarrite tradizioni e legami secolari. Nella sua azione, la Regione Umbria ha perso di vista la persona, la famiglia, le radici, le tante comunità presenti sul territorio. Per chi non lo sapesse, solo qualche mese fa, dopo 12 anni, un'intera comunità di baraccati è stata evacuata da una sistemazione ormai igienicamente insostenibile

ma certo, ciò potrà avvenire se resterà alta l'attenzione dell'intero Paese, se i terremotati non saranno lasciati soli. Quando ho saputo che il G8 si terrà all'Aquila, all'Aquila, che il Consiglio dei ministri si è riunito più volte proprio nelle zone terremotate, ho toccato con mano questo nuovo modo di affrontare i problemi, un modo che farà scuola per il futuro a

sono stati colpiti da una catastrofe naturale di vaste proporzioni. Ci siamo sentiti uniti, davvero tutti uniti, e nel momento del pericolo abbiamo ritrovato una solidarietà profonda. Nel merito del provvedimento, voglio sottolineare la mole imponente delle risorse stanziate, pari a circa 8,5 miliardi di euro complessivi, di cui 1,5 miliardi di euro per l'immediato.

Signor Presidente, onorevoli senatori, rappresentante del Governo, gli eventi sismici che hanno colpito la Regione Abruzzo, con una serie di scosse consecutive a partire dal 6 aprile scorso, rappresentano senz'altro un evento catastrofico dalle dimensioni disastrose, cui il Governo ha fatto fronte prontamente con una serie di ordinanze della protezione civile e con il decreto‑legge in esame, stanziando i finanziamenti necessari per uscire dall'emergenza. Il decreto-legge ha ricevuto una serie di critiche da parte degli enti locali interessati e degli operatori economici e, soprattutto, da parte dell'opposizione durante l'esame del provvedimento in Commissione, come per altro dimostra il cospicuo numero di emendamenti presentati - circa 630

Vorrei tuttavia denunciare la mancata soluzione di uno dei punti critici, che è importantissimo perché comporta conseguenze negative e immediate sull'intero Paese. Si tratta del comma 5 dell'articolo 14, che, ai fini del recupero di risorse finanziarie, revoca i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti prima del 31 dicembre 2005, qualora gli enti locali mutuatari non abbiano provveduto a richiedere il versamento almeno parziale. Si tratta di mutui concessi sulla base di leggi speciali, che prevedono l'ammortamento a totale carico dello Stato. La disposizione è senz'altro utile per recuperare i fondi di vecchi progetti abbandonati dalle amministrazioni o anche, si potrebbe dire, per «punire» quegli enti locali che, per inerzia e inadempienza, non sono stati in grado di spendere le risorse appositamente messe a disposizione dallo Stato. Ma la formulazione del testo penalizza anche quei Comuni che hanno registrato ritardi provocati non da una loro colpa, ma da sopravvenute modifiche dei progetti delle opere o da sopraggiunte esigenze di conversione di scelte operative, dettate magari dal progresso della tecnologia; scelte che, vista l'assegnazione centralizzata delle risorse, sono state magari decise di concerto con il Ministero delle infrastrutture spesso le lentezze amministrative dei Ministeri hanno bloccato l'approvazione dei progetti e hanno impedito ai Comuni beneficiari dei finanziamenti di accedere ai mutui. Ritengo che tali situazioni debbano essere escluse dalle penalizzazioni conseguenti all'applicazione del comma 5 dell'articolo 14. Giusto per fare un esempio concreto, cito il progetto della tramvia di Verona, approvato dal CIPE con un finanziamento pari a 124 milioni di euro per il primo lotto funzionale. Il progetto è stato successivamente modificato, in accordo con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e trasformato in un sistema filoviario che permette il raddoppio dei chilometri di linea (che passano da 10 a 24), con un minore costo per lo Stato dell'ordine di 84 milioni di euro. La documentazione di progetto è stata firmata alcuni giorni fa dal ministro Matteoli ed è stata inviata al CIPE per l'approvazione. Ovviamente, in attesa dell'approvazione del CIPE, il Comune non ha ancora potuto richiedere il versamento del mutuo. Sembra che altri progetti si trovino in situazioni analoghe. Un primo elenco dei Comuni interessati include le metropolitane e tramvie di Latina, Napoli, Palermo, Firenze e Genova. Il mio Gruppo ha presentato una serie di emendamenti tesi a risolvere le incongruenze della norma, oltre che a sopprimere l'intero comma 5, che sembrerebbe la soluzione più desiderata da tutti. Il primo emendamento esclude dalla revoca i mutui relativi a interventi oggetto di modifiche progettuali o di conversione di scelte operative, per i quali sono in corso le relative istruttorie di approvazione da parte del CIPE. Il secondo emendamento prevede invece la revoca dei mutui attraverso un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare sentite le competenti Commissioni parlamentari, previa ricognizione della mancata persistenza di interesse per la realizzazione delle opere. Altri emendamenti trasformano la revoca dei mutui in "sospensione" permettendo nell'immediato l'utilizzo temporaneo delle risorse per l'emergenza terremoto. Peraltro, visto che si tratta di opere approvate con leggi speciali, e quindi con leggi che sono state approvate dalle Assemblee parlamentari e non da decreti ministeriali attuativi di norme delegate, riteniamo giusto che il Parlamento possa dire la sua su un eventuale definanziamento di tali opere. Indipendentemente dall'approvazione o meno dei nostri emendamenti, chiediamo pertanto al Governo di intervenire prontamente per risolvere la situazione, evitando di definanziare opere importantissime per i trasporti delle maggiori città del Paese. Un altro punto su cui mi vorrei soffermare riguarda l'eccellente lavoro svolto dal volontariato in questa straordinaria situazione di emergenza terremoto. I dati forniti dal Governo evidenziano più di 10.000 soccorritori, 5.473 tende, distribuite in ben 169 aree di ricovero, 100 cucine da campo, 3.600 bagni. In questa distribuzione di servizi, il lavoro del volontariato è stato consistente e importante. Ma occorre fare una considerazione sul volontariato, mettendosi anche dalla parte degli imprenditori e degli artigiani che, specialmente nell'occasione del terremoto dell'Abruzzo, hanno visto svuotate le proprie aziende del personale arruolato alla protezione civile. Ovviamente i volontari dipendenti devono avere il proprio stipendio dal loro datore di lavoro, somme che l'imprenditore recupera dallo Stato con una giusta, ma interminabile burocrazia che purtroppo oggi dura circa 2 anni. Vista l'attuale crisi economica tali costi si rivelano assai elevati per le piccole aziende e per i piccoli artigiani. Anche in considerazione dell'ammontare delle persone impegnate nel terremoto dell'Abruzzo, spesso diventa molto oneroso per le aziende poter pagare comunque i dipendenti, anche se questi ultimi mancano dal lavoro perché impegnati in attività della protezione civile. Pertanto, con un nostro emendamento abbiamo previsto la possibilità per i datori di lavoro di persone impegnate nel volontariato di compensare nel modello F24 i rimborsi che devono avere dallo Stato per gli emolumenti anticipati. Mi auguro che quest'Aula e il Governo

dell'ampliamento della fascia dei benefici, anche se è estremamente importante - me ne rendo conto - che i

le stesse istituzioni dello Stato hanno sollevato il problema del danneggiamento di una serie di edifici pubblici e privati - mi riferisco tra

Gran parte del provvedimento è destinata ad accompagnare le vicende singole e familiari delle persone colpite dal terremoto nelle articolazioni

eccezione fatta per quelli che rivestono particolare urgenza. L'articolo 6 regola i comportamenti dell'amministrazione, prevede

le deroghe previste per il personale di sicurezza e per il personale di protezione civile e l'ampliamento delle provvidenze ai lavoratori, in maniera tale che nessuno si senta escluso e che quindi la coesione sociale non sia messa in discussione da un evento drammatico come quello sismico di cui stiamo parlando.

deve comunque esserci una copertura da parte dello Stato. Sostanzialmente si stabiliscono dei principi e un ampliamento della sfera delle provvidenze, in maniera tale da rassicurare e dare speranze di una ripresa, assistita e agevolata dallo Stato, a tutta la popolazione. Nello stesso tempo, con una una declaratoria della tipologia degli interventi che si intende favorire, si avvia la fase della ricostruzione.

si favoriscono dei provvedimenti di urgenza e quindi si accettano delle deroghe, con un giusto equilibrio, a mio parere,

che consentano di accelerare le procedure di localizzazione e quindi di ricostruzione, tenendo conto che si tratta di comuni montani e che quindi in molti casi si deve procedere con una rapidità ancora maggiore rispetto a situazioni meno disagiate dal punto di vista atmosferico.

chiede un aiuto organizzativo per garantire il sostegno e il supporto all'attività di ricostruzione; che deve essere accompagnata da criteri di sicurezza, non soltanto dal punto di vista della tecnica ricostruttiva, dell'antisismicità

l'organismo centrale ministeriale presso la prefettura dell'Aquila, un particolare servizio di monitoraggio e di attenzione nei confronti del pericolo della partecipazione della criminalità organizzata alla ricostruzione. Infine, non si può non citare lo

menzione di solidarietà e di qualità nello stesso tempo, del provvedimento. È una testimonianza del fatto che non soltanto vicino a chi in quel momento ha più bisogno e più soffre, ma è una testimonianza (anche per come è stata vissuta dalla regione Sardegna, che va per dello Stato. È un bell'esempio di esistenza in vita dello Stato stesso, perché senza questo concetto di solidarietà viene a mancare lo stesso concetto di esistenza in vita dello Stato. Mi piaceva quindi rimarcare questi aspetti del provvedimento, che ritengo qualitativamente di grande livello.

non sono aduso a fare il processo alle intenzioni e, quindi, mi guardo bene dall'affermare che dietro lo spostamento del G8 dalla Sardegna all'Abruzzo possa esserci soltanto il tentativo di esercitare una cinica mossa a sorpresa per costruire consenso lucrando sulle disgrazie altrui. Voglio evitare di rendere questa affermazione per evitare di commettere eventualmente un errore. Voglio però cercare di commentare alcuni fatti concreti riguardanti la terra di Sardegna la quale, come appena ricordato dal collega Cicolani, è una terra che in moltissime circostanze ha direttamente e concretamente manifestato la propria solidarietà. Signor Presidente e cari colleghi, diversamente da quanto normalmente succede allorché in un Paese - parliamo del nostro - si realizza un appuntamento di carattere internazionale quale il G8,

È stato detto stamattina da un autorevole collega della maggioranza, riferendosi alla Sardegna, che il Premier avrebbe esercitato un'azione incisiva e che in Sardegna tutti sarebbero contenti. L'incisività dell'azione del Premier, signor Presidente, purtroppo si è sviluppata a danno dei sardi. Dopo aver attraversato in lungo e largo, per almeno cinque fine settimana, il nostro territorio regionale in occasione della campagna in occasione della campagna elettorale per la Regione Sardegna, per sostenere e magnificare la straordinarietà dell'evento e la volontà del Premier in prima persona di renderlo strumento particolarmente utile per risarcire l'Arcipelago della Maddalena per i trent'anni di asservimento agli interessi internazionali, con i sottomarini a testata nucleare nelle acque territoriali, e un'intera isola

questo, il presidente ha ritenuto, *motu proprio*, senza neanche comunicarlo al presidente della Giunta regionale, di presentare un provvedimento per cancellare tutto.

Il Gruppo del Partito Democratico ha presentato una serie di emendamenti all'articolo 17, perché quantomeno si faccia giustizia; perché la solidarietà, che deve essere ben altro rispetto a quanto contenuto nel decreto che stiamo discutendo, si esprima copiosa, significativa e sincera a beneficio della sfortunata popolazione abruzzese, ma senza che ciò si verifichi a danno dei sardi: sono stati cancellati appuntamenti internazionali; sono state cancellate strade che avrebbero dovuto unire gran parte di una Sardegna priva di infrastrutture; sono stati cancellati interventi di carattere igienico-sanitario. E il tutto è stato fatto vergognosamente, dopo aver saccheggiato a piene mani la buona fede e la stessa dignità dei sardi. Se è rimasto un sussulto di sensibilità e - me lo lasci dire - anche di dignità nei confronti di una terra che non vuole più pacche sulle spalle, sorrisi gratuiti, ma fatti, c'è l'opportunità di approvare i nostri emendamenti. Diversamente, si abbia almeno il buon gusto di smetterla con questa terribile presa in giro.

di tutta la macchina amministrativa della Regione, della Provincia, del Comune capoluogo, di tutti gli enti e le istituzioni ivi presenti, dal tribunale alla sede dell'ANAS, dalla struttura della Protezione civile stessa

non si potevano attendere, come in passato, tre, quattro, cinque o otto mesi per avere il primo decreto e nel frattempo andare avanti con la provvisorietà, perché purtroppo

non abbiamo ancora la precipua contezza di quale sia effettivamente il danno, di quali siano le effettive esigenze e le risorse necessarie per pensare ad una completa ricostruzione, non soltanto della struttura urbana

È evidente che questa Camera, come l'altra ed il Governo tutto, dovranno ancora, purtroppo per molti mesi, tenere sulla loro agenda la questione abruzzese e noi parlamentari abruzzesi saremo in prima linea a ricordarlo, se mai ce ne fosse bisogno.

necessaria alla ricostruzione e alla rinascita di un territorio colpito dal terremoto. Apprezziamo la vicinanza e l'affetto dimostratici da tutti quanti i senatori presenti,

e che si sia dissipata ogni nebbia, perché sulla prima casa l'articolato parla chiaramente di un rimborso al cento per cento con un fondo speciale e con un finanziamento a fondo perduto.

altro provvedimento fondamentale richiesto dal territorio e che ha trovato riscontro proprio nell'accoglimento da parte del Governo degli emendamenti proposti in Commissione. Se questo e altri punti sono significativi per testimoniare il buon lavoro svolto in Commissione e le ulteriori migliorie apportate al testo, che già di per sé era apprezzabile, credo però senza punta di polemica mi si possa permettere di non accettare che qualche collega di opposizione, in particolare modo il collega Lusi,

che testimoniano la nostra presenza maggioritaria qui dentro vorrebbero dire che responsabilità e meriti appartengono a una sola parte politica. Credo invece che il senso di responsabilità di tutti noi ci debba far dire che, se è vero che questo provvedimento

che certamente non è conclusa l'attenzione del Governo e delle Aule parlamentari al terribile terremoto che ha colpito la nostra Regione. Dovremo tornare ancora tante altre volte su questo argomento, e per tanti molteplici aspetti, perché una volta superato il tema della ricostruzione - e penso che con questo decreto

altre saranno le priorità che dovremo contemperare in passaggi successivi, con provvedimenti normativi ma anche con sedute apposite. apposite. Penso in particolare ad un passaggio che dovremo necessariamente approfondire anche in questa sede, quello per cui questo terremoto verrà purtroppo tragicamente ricordato: il crollo della Casa dello studente e la situazione del nosocomio San Salvatore. Dovremmo chiederci anche se ci sono state e vi sono responsabilità,

che questo provvedimento, che è stato straordinario dal punto di vista della celerità,

purtroppo sono ancora sul tappeto della Regione Abruzzo e, conseguentemente, sul tavolo del Governo. Signor Presidente, come i colleghi avranno avuto modo di rilevare, la discussione è estremamente interessante ma anche estremamente collaborativa da parte di tutti colleghi. Vorrei quindi brevemente utilizzare

abbia sottolineato l'importanza della normativa antisismica, che in Commissione abbiamo affrontato anche intervenendo sulla revoca della proroga, decisa nel corso dell'ultimo decreto milleproroghe, ai fini dell'attuazione della normativa antisismica sul territorio nazionale. Anche i suoi interventi sulla *governance* sono già stati oggetto di discussione in Commissione. Ho avuto più volte maniera di sottolineare come, a mio giudizio, si possa certamente ampliare il tema della *governance* mediante il coinvolgimento degli enti locali nella fase della ricostruzione e

quindi con un accordo di fatto. È chiaro che la norma deve proteggere un *iter* operativo che ha tempi ristrettissimi, assolutamente improrogabili e cadenzati,

ha in mente di escludere le competenze degli enti locali; anche nell'intervento del senatore Monti abbiamo apprezzato questo richiamo: è nel DNA di ognuno di noi, soprattutto di coloro che hanno avuto esperienze amministrative locali, tenere nella massima considerazione l'apporto costruttivo che gli enti locali possono dare, anche in un regime di emergenza e d'urgenza come quello che ci troviamo ad affrontare. Da questo punto di vista mi sento di condividere le valutazioni del senatore Fleres, che ha parlato della necessità di un quadro a regime per la protezione civile e, soprattutto, per la prevenzione.

Il Parlamento quindi dovrà prendere in considerazione norme di più ampio respiro, che possano cominciare a segnare nel nostro Paese una vera politica della prevenzione

la ricostruzione e gli indennizzi per sanare le ferite del territorio costi molto più di quanto non possa costare l'intervento di prevenzione costare l'intervento di prevenzione che, se adeguatamente strutturato sul territorio, può anche consentire l'accesso a strumenti di negoziazione privata come, ad esempio, le assicurazioni, che possono tranquillizzare tranquillizzare il cittadino e mettere lo Stato ed il Governo nelle condizioni di intervenire in maniera

ad ampliare quanto più possibile le norme relative alla prevenzione, a sollecitarne l'utilizzo ed a superare le perplessità - come le cronache di questi giorni hanno riportato - provenienti dagli stessi enti locali, dalle stesse autonomie locali.

i dubbi sulla efficacia delle coperture, perché una cosa è l'ammortamento nel lungo periodo da parte del Governo degli oneri che si va ad assumere, altra l'immediata disponibilità che il Governo garantisce. Se poi questa disponibilità viene ammortata, per esigenze di bilancio, in un lungo arco temporale, credo che questo sia assolutamente compatibile con le esigenze del territorio. Con un esempio che può apparire pedestre, caso di un cittadino che volendo acquistare una casa ma non avendone la possibilità, stipula un mutuo ed ottiene l'immediata disponibilità delle somme che pagherà nel tempo contrattualmente previsto. senatore Lannutti - e credo che il Governo ne debba assolutamente fare tesoro - di un atteggiamento estremamente penalizzante degli istituti di credito sul territorio abruzzese, atteggiamento che non ha motivazioni.

che ciò non accadrà o, nel caso sia già accaduto, che verrà immediatamente censurato. Il senatore Pastore ha parlato giustamente di collasso istituzionale delle strutture della Regione Abruzzo,

e resoconti, della grande volontà della città di continuare, anche in condizioni di disagio, ad assolvere al suo ruolo istituzionale di Capoluogo di Regione. Da questo provvedimento tale volontà deve uscire

degli interventi del Governo, sia sulla correttezza delle valutazioni in ordine alla copertura, sia sulla capienza del Fondo indicato dall'articolo 14 al comma 1. 1. Il problema della zona franca urbana lo abbiamo trattato in Commissione, e con questo faccio riferimento non solo all'intervento del senatore Tancredi ma a tutta una serie di interventi che sono stati fatti in Aula. La zona franca urbana, che è stata approvata in Commissione con un emendamento del relatore che nasceva dalla comune volontà delle forze politiche, è certamente un rimedio importante per rivitalizzare immediatamente l'economia dei territori disastrati. Vi è anche un emendamento da me presentato perché le provvidenze relative alla zona franca urbana, approvate in Commissione con riferimento al solo anno 2009, vengano estese agli anni 2010 e 2011 con un eguale stanziamento di 45 milioni di euro per ogni anno. anche con una certa preoccupazione quanto riferito dal senatore Astore in ordine allo sciacallaggio e allo svuotamento dell'università dell'Aquila. Non per nulla

su questo il Governo avrà maniera di intervenire; così come - lo ribadisco - nell'ambito di questo provvedimento la tutela delle attività didattiche, a livello non solo universitario, ma anche di istruzione primaria e secondaria, è assicurata da tutta una serie di autorizzazioni al Ministro della pubblica istruzione per intervenire anche con i relativi stanziamenti. Il senatore Lusi poi ha fatto una nota abbastanza dettagliata delle ulteriori problematiche che, a suo giudizio, rimangono da risolvere affinché,

Premetto che, a mio giudizio, già così com'è questo decreto risolve la stragrande maggioranza dei problemi immediati dell'Abruzzo e che, come più volte ci ci si è detti, questo non può essere l'unico provvedimento che interviene in favore delle popolazioni abruzzesi. La tematica è in continuo divenire; le rilevazioni sul territorio non sono ancora state conosciamo con esattezza, anche se ormai il *trend* statistico ci dice che le abitazioni che saranno rioccupabili a breve dagli abitanti dell'Abruzzo superano di di buona misura il 50 per cento del patrimonio immobiliare della stessa Regione e delle zone colpite. Anche se, lo ripeto, abbiamo rilevazioni ogni giorno sempre più confortanti sulla possibilità di intervenire rapidamente per risanare almeno per il 70 per cento l'intero patrimonio abitativo delle zone terremotate, credo che non mancherà la necessità

l'esigenza dell'emergenza, ma anche dei tempi brevi), dà la possibilità al Governo di completare gli interventi attraverso l'emanazione di successive ordinanze, come

spesa di ricostruzione, riattamento o riacquisto - a seconda di quanto venga deciso dall'interessato - per le case dell'abitazione principale. certamente già un elemento di chiarezza importante. La residenzialità viene quindi assicurata nella ricostruzione attraverso questa certezza, così come abbiamo chiarito

del credito d'imposta che, da un ulteriore chiarimento che viene dal Governo, può essere utilizzato anche per il pagamento delle rate dei finanziamenti agevolati cui fa riferimento l'articolo 3

parte delle richieste, che anche oggi sono state illustrate nel corso di una conferenza stampa dal Partito Democratico, siano già contenute

mantenere vigile lo sguardo, soprattutto per continuare a catalizzare eventuali risorse che possono venire dalla solidarietà internazionale. È giusto anche alle imprese locali, alle loro possibilità di ripresa, all'opportunità di sostenerle in questo momento di difficoltà con riferimento alla commercializzazione dei propri

sottolineato alcune criticità riguardanti la norma sulla Cassa depositi e prestiti. Ritengo che il Governo interverrà a chiarimento di quelle che sono le effettive conseguenze di questa norma che intende, non solamente fare cassa (è chiaro, però, che è utile anche per la cassa), ma, soprattutto,

che è indirizzato soprattutto ad evitare che risorse disponibili giacciano nella insipienza delle amministrazioni locali perché non adeguatamente utilizzate. Allo stesso tempo, le amministrazioni che stanno utilmente attivando quelle norme saranno sicuramente protette e confermate dalle procedure ministeriali necessarie. Il senatore Cicolani ha sottolineato come sia assolutamente innovativo il carattere del decreto-legge, non solamente per quanto riguarda l'impianto normativo delle ordinanze e della legge (ossia del combinato disposto tra ordinanza e legge), ma soprattutto con che, per la prima volta, sono orientati, non solamente alla ricostruzione fisica dei luoghi, ma anche ad accompagnare le popolazioni dell'Abruzzo verso la ripresa socio-economica. L'attenzione alle strutture L'attenzione alle strutture (anche produttive), ma soprattutto ai comparti produttivi e ai lavoratori (grazie alle norme che prevedono interventi straordinari di cautela dei lavoratori e interventi - penso, per esempio, al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

sono stati assolutamente collaborativi in termini di proposte e tutti hanno invariabilmente riconosciuto l'efficienza e l'efficacia dei primi interventi della Protezione civile e del Governo, nonché l'impegno l'impegno che il Presidente del Consiglio ha personalmente dispiegato nella sua attenzione per le popolazioni dei territori devastati dal sisma e la volontà che l'impegno, l'efficienza e l'efficacia dei primi momenti possano essere consolidati

In ultimo, credo che non sia inutile sottolineare come quasi tutti abbiano speso parole di sollecito per l'intervento sui beni culturali dell'Abruzzo: l'ho fatto anche io nel corso della mia relazione, ma soprattutto lo ha fatto la Commissione attraverso l'approvazione di alcuni emendamenti. Siamo tutti convinti - e certamente il Governo, per come ci dirà, ne è consapevole che nelle terre devastate dal terremoto (non solamente dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista morale e delle testimonianze autentiche della nostra civiltà) gran lì conservato, sia stato oltraggiato dall'evento sismico e sia da recuperare nella sua interezza e con oneri a carico della collettività nazionale. Infatti, non è patrimonio di quelle terre, ma è patrimonio dell'intera

è un importante passo parlamentare nel quale è giusto e doveroso si vivano momenti alti di solidarietà nazionale.

Ciò ha dimostrato come anche queste Aule non siano solo quello che spesso banalmente si dice, cioè luogo di teatro, di tribune e di scontro politico, ma anche luoghi e momenti

Il terremoto che il 6 aprile scorso ha devastato l'Abruzzo ha visto una pronta risposta non solo da parte dell'apparato statale, ma anche di tutto quello che rappresenta il mondo del volontariato di tutto quanto è stato in grado di organizzare la nostra Protezione civile. Anche sotto questo profilo, con un pizzico di orgoglio, devo dire che anche in momenti drammatici come questi l'Italia dimostra di avere sempre un qualcosa in più,

impostato su un impianto normativo e procedurale già sperimentato, peraltro, con successo in occasione di altri eventi calamitosi, che si articola sostanzialmente in due fasi.

che consentano l'avvio di interventi urgenti. Siamo nella fase della prima emergenza, quella cosiddetta straordinaria.

la fase, ancora più importante, della ricostruzione, che individua, com'è doveroso, le fonti di copertura e mantiene sempre il riferimento allo strumento dell'ordinanza, proprio perché esso è particolarmente agile e flessibile - dato che si opera in una situazione fuori dall'ordinario - e consente comunque aggiustamenti in corso d'opera e di relazionarsi con il fatto così come accade, anche non prevedibile. È infatti del tutto evidente è difficile normare tutto ciò che non è prevedibile. Allora si può agire in un contesto generale di norma; poi però è inevitabile servirsi dell'ordinanza nel concreto. Per cui una serie di fatti e di atti vengono compiuti a seguito e sotto l'ombrello del decreto-legge, che diventerà poi legge, ma passano attraverso questo diverso strumento. La fase straordinaria si è conclusa - purtroppo dovendo contare 298 uomini e donne da piangere da piangere - con l'allestimento immediato di una struttura che ha messo in campo una capacità di risposta alla domanda di allocazione di 65.000 persone.

ha deciso di fare? Più di qualcuno in quest'Aula ha fatto notare come L'Aquila sia una città particolarissima dove, come si diceva, l'inverno finisce dopo ma inizia prima. prima. Noi siamo pienamente coscienti che ad ottobre dovremo essere in grado di dare davvero una casa

40.758 edifici, divisi tra privati, pubblici, ospedali, scuole, caserme e attività produttive

Ciò vuol dire che, in tempo breve, due persone su tre potranno sostanzialmente ritornare a casa. Il 2,9 per cento degli edifici risulta parzialmente inagibile,

riprendendo la dizione del decreto, contempla la realizzazione di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, nonché delle opere connesse di urbanizzazione, com'è ovvio. Tali moduli abitativi sono immediatamente destinati a consentire la più sollecita sistemazione delle persone le cui abitazioni sono distrutte e inagibili. Tali abitazioni, oltre al rispetto di tutte le norme di sicurezza socio-sanitarie, devono anche rispondere ad una serie di caratteristiche che abbiamo formalmente individuato: elevati livelli di qualità, innovazione tecnologica orientata all'autosufficienza impiantistica e protezione sismica anche mediante isolamento sismico per interi complessi abitativi. Questo significa che gli edifici verranno posati

di ulteriori fasi sismiche. Come è noto, ad un sisma di notevole intensità, quale quello avvenuto, segue sempre uno sciame sismico che non necessariamente è decrescente potendo ritrovare delle punte.

la Commissione non approva un testo diverso ma sostanzialmente lo propone, quindi non si arriva in Aula con un testo proposto dalla Commissione, come avviene alla Camera (quel Regolamento lo conosco bene, questo di meno, lo devo imparare). il Governo si è fatto promotore di un emendamento che ha risposto alla prima grande questione che era stata posta, vale a dire: il contributo copre integralmento o no la casa perita, caduta, distrutta?

Non solo, nel testo originario rimaneva una difficoltà interpretativa paradossale, perché si poteva intendere che abitazioni solo danneggiate ma non dichiarate inagibili non fossero coperte dal contributo. La questione è stata chiarita nello stesso emendamento. Sono abituato alla Camera, dove c'è ancora più rumore, di solito.

la concessione del contributo stesso anche con la modalità di credito d'imposta o di finanziamento agevolato - ha chiarito che il contributo, di cui all'articolo 3, è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di alloggio equivalente. Come pure è specificato

la prima volta ci si è trovati di fronte ad un terremoto che ha colpito una città capoluogo di Regione e a così alta densità di patrimonio artistico e storico. di vista, il Governo è pienamente cosciente della ricchezza artistica dell'Aquila, che rende sicuramente più difficile la ricostruzione, soprattutto per quei per quei particolari edifici vincolati o comunque individuati come di interesse artistico (parliamo di monumenti storici, di musei, di chiese, ma anche di abitazioni private), tant'è che da una prima stima al riguardo risulta che almeno 400 milioni di euro sono da destinare immediatamente ai beni artistici.

È quindi assoluta intenzione del Governo rispondere con fatti concreti a tutto questo, riaffermando la centralità dell'Aquila all'interno della Regione Abruzzo, rendendo funzionali

Ed è proprio su questa scommessa per il futuro che si innesta - anche se riguardo ad una questione parzialmente diversa - un altro tema del dibattito che si è svolto, tanto in Commissione, quanto oggi in Aula: quello che concerne la *governance* dell'opera di ricostruzione.

2, piani di ricostruzione del centro storico delle città definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica e la riqualificazione dell'abitato, nonché per facilitare il rientro delle popolazioni sfollate nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici. Questi erano sostanzialmente i punti nodali del dibattito che si è svolto e credo che vi sia stata una risposta positiva; non tutto è chiuso (è evidente), però mi pare che, nella corretta dinamica del rapporto tra Governo, maggioranza e opposizione, molto si sia costruito.

la realizzazione delle abitazioni, le agevolazioni per la ricostruzione, gli indennizzi a favore delle imprese e la ricostruzione degli uffici pubblici. Vi sono poi norme di contorno che provvedono a normare la situazione emergenziale di oggi: si pensi per esempio a tutta la questione della sospensione dei termini,

puntualizzato bene la questione del Patto di stabilità: è evidente che sono fuori dal Patto di stabilità gli interventi fatti in conseguenza dell'emergenza. Vi è la previsione di una serie di provvidenze in favore delle persone fisiche e delle imprese;

si deve creare un sistema di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali derivanti dal crollo; vi sono disposizioni intese ad agevolare lo sviluppo economico e sociale; vi sono altre disposizioni che qualcuno definisce aleatorie, ma io penso che tutto l'articolo 12 - per capirci, quello dedicato ai giochi - dia comunque una serie di garanzie anche in termini di aggiunta alla copertura; vi sono disposizioni che riguardano la spesa farmaceutica; vi sono misure di carattere finanziario; anche un'attenzione, che ritengo assolutamente utile e condivisa sicuramente da ogni fronte di quest'Assemblea, per cui al prefetto dell'Aquila è delegato il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata che, com'è noto, in situazioni di questo genere ci sguazza o tenta di farlo;

all'Aquila non è una sorta di *show*, perché non si viene a vedere uno spettacolo che ad uno *show* potrebbe essere paragonato, quanto piuttosto mi pare segno di attenzione che serve anche a fortificare la solidarietà internazionale nei nostri confronti.

sappia trarre tutto ciò che di positivo si può trarre dalla discussione e dal dibattito, migliorando il testo di questo decreto. Ripeto, già molto è stato fatto in sede di Commissione e non dubito che ciò avverrà anche in Aula.

luttuosi che talvolta lo colpiscono, sa mostrare una solidarietà è un'umanità che in altri luoghi è sconosciuta. Grazie, signor Sottosegretario, anche per lo sforzo che ha fatto in condizioni non ottimali di ascolto.

di cittadini; l'A.S. 1534 (Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile) prevede, 1a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, nel presupposto che il decreto-legge contiene norme di carattere eccezionale e speciale in ragione della straordinaria gravità degli eventi che sono specificamente indicati all'articolo 1, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni: all'articolo 2, comma 8, appare necessario prevedere che i provvedimenti del Commissario delegato siano adottati previa consultazione del Presidente della Regione Abruzzo; - all'articolo 4, occorre tenere conto delle competenze delle Regioni e degli enti locali per la fase di attuazione della ricostruzione. Esaminati altresì gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri: - sugli emendamenti 1.300 e 2.300, parere non ostativo, a condizione che, in luogo dell'intesa tra gli enti locali interessati, sia disposta la semplice acquisizione del parere, al fine di evitare il rischio di arresto dei procedimenti ivi previsti; sull'emendamento 2.12, parere contrario, in quanto la norma determina una violazione delle competenze costituzionalmente attribuite alle Regioni e agli enti locali; - sull'emendamento 2.302, parere non ostativo, osservando che la soluzione ivi configurata, rispetto a quanto contenuto nel testo, sembra ridimensionare il coinvolgimento degli enti locali, dal momento che, in luogo del parere di un'apposita conferenza di servizi, prevede il parere della sola provincia dell'Aquila; - sull'emendamento 3.0.9, parere non ostativo, a condizione che siano salvaguardate le competenze dei Comuni in materia di urbanistica; sull'emendamento 4.726, parere non ostativo, nel presupposto che siano chiariti gli strumenti di intervento sostitutivo del Ministero del lavoro, della salute e della politiche sociali, al fine di evitare possibili sovrapposizioni di competenze con la Regione; sull'emendamento 4.319, parere non ostativo, nel presupposto che sia garantita la competenza dell'ente Regione nell'assegnazione delle risorse alle aziende sanitarie locali; - sull'emendamento 4.323, parere non ostativo, rilevando l'opportunità di chiarire cosa si intenda per "comitato di affiancamento" e quali debbano essere le sue funzioni; - sull'emendamento 6.718, parere non ostativo, a condizione che, al capoverso 4-*bis*, siano configurati come facoltà, e non come obblighi, i compiti ivi attribuiti al Comune e alla provincia dell'Aquila; sull'emendamento 10.0.1, parere contrario, per violazione dell'articolo 117, sesto comma della Costituzione, che attribuisce allo Stato la potestà regolamentare solo nelle materie di legislazione esclusiva,

sull'emendamento 12.8, parere non ostativo, segnalando la possibile compressione delle competenze delle Regioni e degli enti locali in riferimento ai compiti della polizia municipale; - sui restanti emendamenti parere non ostativo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo reso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti condizioni: che all'articolo 2, comma 13, le parole «dal comma 10» siano sostituite dalle seguenti: «dai commi 10 e 12»; - che all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, siano espunte le parole: «escluse le procedure di esecuzione coattiva tributaria»; che all'articolo 6, dopo il comma 3, sia inserito il seguente 3-*bis:* «Le misure di cui al comma 1, lettera da *a)* ad *n)* della presente disposizione, possano essere attuate limitatamente all'esercizio finanziario 2009, nell'ambito delle risorse di cui al comma 4»; che all'articolo 7, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «Corpo nazionale dei vigili del fuoco» siano inserite le seguenti: «; a tal fine è autorizzata la spesa di 1,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009»; che all'articolo 12, comma 2, venga in fine aggiunto il seguente comma: «2-*bis.* All'attuazione delle norme di cui al comma 2, si deve provvedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tal fine, il personale trasferito mantiene il trattamento economico in godimento»; che all'articolo 13, comma 1, lettera *a),* quarto periodo, dopo le parole: «è effettuata» vengano introdotte le altre: «nell'anno 2009»; - che al comma 6 dell'articolo 16 venga aggiunto in fine il seguente periodo: «Resta fermo che il Ministero dell'interno provvede al conseguimento dei risparmi di spesa previsti dal comma 416 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 mediante la razionalizzazione delle rimanenti articolazioni del ministero medesimo». Il parere è altresì reso con i seguenti presupposti: - che, in ordine all'articolo 6, comma 1, lettere *o)* e *p),* in relazione alla deroga al Patto di stabilità interno, siano utilizzate dagli enti interessati le sole risorse previste dal provvedimento; che, in ordine all'articolo 6, comma 1, lettera *r),* la fattispecie non si riferisca a sanzioni già accertate; - che in relazione all'articolo 8, lettere *a), b)* e *c),* siano rispettati i vincoli temporali indicati nella relazione tecnica assunti a fondamento delle relative stime».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi agli articoli da 1 a 3 del disegno di legge in titolo trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.600/1, 1.6, 1.7, 1.16 1.22, 1.23, 1.30, 2.54, 2.55, 3.18, 3.20, 3.28, 3.0.7, 3.0.7, 1.306, 1.307 e 3.0.302. In ordine alla proposta 1.705, il parere è non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla previsione che l'operato dei componenti degli organi previsti sia a titolo gratuito. In ordine alla proposta 2.312, il parere è non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria nonché alla previsione che non spettino compensi ai componenti dell'organo istituzionale. In ordine alle proposte 3.307 e 3.0.300, il parere è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria. In ordine alle proposte 3.307 e 3.0.300, il parere è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria. In ordine alla proposta 3.0.301, il parere è non ostativo, reso alle seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: - che sia inserita una clausola d'invarianza finanziaria; - che al comma 2, secondo periodo, siano espunte le parole: ", nonché alle ulteriori agevolazioni fiscali e contributive necessarie in relazione agli effetti dannosi dell'evento". Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti fino all'articolo 3, ad eccezione che sulle proposte 2.800 e 3.5000, sulle quali l'espressione del parere è sospesa».

il mio parere è contrario, considerando che, in ogni caso, così com'è non potrebbe essere accolto perché ogni suo punto dovrebbe essere oggetto di approfondimento e di dibattito.

ogni caso, ripeto, la seconda parte del dispositivo, a mio giudizio, dovrebbe essere ritirata e la prima parte dovrebbe essere preceduta dalle parole: «a valutare l'opportunità di prevedere».

Forse è più semplice che io lo legga come ritengo che debba essere formulato: «...a valutare l'opportunità di prevedere l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta per consumi di gas metano per uso promiscuo, nonché l'applicazione di un'aliquota IVA agevolata per consumi di gas metano per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda». Questa mi sembra una formulazione più idonea ad un ordine del giorno, poi valuti il Governo se debba accoglierlo o meno: a mio avviso, potrebbe essere accolto come raccomandazione.

G10, della Commissione, riguarda lo sforzo per garantire la ripresa immediata delle attività didattiche: nato da un ordine del giorno presentato dalla senatrice Soliani, è stato accolto dalla Commissione, quindi ne raccomando l'accoglimento al Governo.

trattandosi della vera e propria scrittura di una proposta normativa in ordine ad una risistemazione dell'intero patrimonio immobiliare nazionale:

del Governo e segnatamente del Ministero della giustizia valutare l'opportunità di questa previsione, inserirei nel dispositivo le parole «a valutare l'opportunità

notazione di impostazione letterale del provvedimento, mentre sarebbe più opportuno che su quest'ordine del giorno esprimesse il parere un esponente del Ministero della giustizia.

mentre è evidente che il G19 ha una propria finalità, che interviene sulla prevenzione nel senso di apprestamento di strutture idonee ad affrontare eventuali emergenze.

di esse, per le proprie competenze, deve eventualmente ricevere una segnalazione da parte del Governo centrale, valutando l'opportunità di alcuni provvedimenti di stabilizzazione - possa avere sempre a disposizione un nucleo efficiente di protezione civile pronto a intervenire in ogni momento

su cui il relatore e il Governo hanno proposto delle riformulazioni che il presentatore accetta. Quindi, le vostre firme riguardano gli ordini del giorno riformulati? le nostre firme, che ho comunicato prima che il primo firmatario dichiarasse la sua disponibilità ad accogliere le richieste del relatore e del Governo, erano e sono sulla versione iniziale degli ordini del giorno.

alla realizzazione di una struttura di protezione civile che non sia precaria e fondata su prestazioni lavorative di tipo precario. Considero in ogni caso un passo in avanti

tra le altre conseguenze del terremoto in Abruzzo, c'è quella, tragica e drammatica, di una sorta di epifania delle questioni le più importanti e le più gravi

il fatto che molte famiglie si siano trovate senza reddito alcuno e senza possibilità di pensare in un futuro prossimo di riprendere il proprio lavoro è certo la rappresentazione esasperata, dovuta al tragico terremoto, di quello che può accadere, ma anche un connotato della fragilità del nostro sistema complessivo di Welfare. Mi riferisco, in particolare, alla questione che riguarda gli ammortizzatori sociali e al fatto che, nonostante alcuni piccolissimi passi avanti siano stati fatti, esistono nel nostro Paese, di fronte alle crisi economiche, che possono intervenire anche per fatti traumatici e radicali come un terremoto, destini di lavoro e umani che vengono consumati senza che vi corrisponda una prospettiva possibile di recupero di un reddito.

che per tutti quei lavoratori che perderanno o hanno già perduto il posto di lavoro e che non sono assistiti dal sistema degli ammortizzatori sociali, così come oggi esiste in questo Paese, siano previste forme altre di estensione di

di non rinunciare alla produzione, ma hanno dovuto per forza ridurre l'orario di lavoro, consegnando così ai loro dipendenti una retribuzione defalcata. Tutto questo ci spinge oggi ed in ragione delle necessità dei lavoratori, delle lavoratrici e delle famiglie d'Abruzzo, e delle difficoltà che incontrano tanti lavoratori e tante lavoratrici italiane, a chiedere un impegno specifico al Governo,

disporre con la massima urgenza, per i prossimi 24 mesi, quindi in misura più generosa e, lasciatemelo dire, più lungimirante di quanto non sia previsto dal decreto, misure misure a sostegno del reddito che siano finalizzate a sostenere le famiglie e gli individui durante questo periodo. Quarto: prevedere un sostegno per i lavoratori che dipendono da imprese, come ricordavo prima, che hanno ridotto l'orario di lavoro.

lavoro. Sesto: fornire finalmente una risposta ai lavoratori e alle lavoratrici d'Abruzzo. Lo dico anche in ragione del fatto che di fronte a tanta diffusione sui mezzi di informazione su ciò che si è fatto in Abruzzo, che ovviamente abbiamo apprezzato nella parte dell'emergenza, restano però sottotraccia una serie di vicende sulle quali forse occorrerebbe riflettere. Per esempio, molti lavoratori delle aziende che fornivano gas ed energia

nell'immediato. Riflettiamo approfittando di questa occasione, perché l'impegno che noi riteniamo essenziale per tutti i lavoratori e le lavoratrici italiane, a partire dai lavoratori d'Abruzzo, sia onorato e per fare in modo che, che, passata la crisi, che ci auguriamo sia a più breve scadenza possibile, l'Italia ritrovi un paese in piedi nella dignità del lavoro e nella dignità di quell'esistenza libera e dignitosa di cui ci parla la Costituzione.

inoltre, il voto favorevole del nostro Gruppo, considerato che uno degli aspetti mancanti nel decreto è la parte relativa alla disciplina del lavoro privato e pubblico

alla scadenza dei rapporti di lavoro precari in alcune importantissime strutture sanitarie dell'Aquila che forniscono un'assistenza delicata e particolare. Noi dobbiamo farci carico anche di tutti questi aspetti, alcuni dei quali sono segnalati (e per questo motivo noi lo condividiamo e sosteniamo) nell'ordine del giorno che ha come prima firmataria la collega Finocchiaro.

C'era stata una disponibilità e una nostra offerta di lavoro comune per utilizzare al meglio il contributo dell'Europa. Quindi, non comprendiamo perché non si potrebbe votarlo tutti quanti.

alla riduzione dell'IVA che con quest'ordine del giorno si invita a valutare,

tra le destinazioni della quota statale le calamità naturali e, visto che stiamo parlando di terremoto e di conservazione dei beni culturali, mi chiedo davvero se in questo luogo le parole abbiano un senso.

la possibilità che sull'ordine del giorno G17, date le competenze specifiche, potesse esprimersi il rappresentante del Ministero della giustizia, ragion per cui mi rimetto al Governo.

il Governo dovrebbe costituire una commissione tecnica, composta da magistrati, personale amministrativo, e quindi da persone che può già utilizzare pertanto ognuno si assume le proprie responsabilità - e questa Commissione tecnica dovrebbe avere il compito di suggerire al Parlamento le attività attività e gli interventi da assumere oppure svolgere attività di raccordo tra soggetti istituzionali (Consiglio superiore, Ministero e dirigenti degli uffici). Credo proprio che l'ordine

raccoglie un invito pressante che ci viene dalla magistratura, dall'avvocatura, dal personale della giustizia abruzzese, a seguito della particolare particolare gravità della situazione che si è venuta a determinare nel settore della giustizia. Com'è noto, non soltanto gli uffici giudiziari dell'Aquila ma anche la Corte d'appello e le magistrature speciali, quali Corte dei conti e e Commissione tributaria regionale, hanno visto determinarsi un blocco totale della loro attività. I fascicoli sono sotto le macerie e vi sono problemi enormi;

delle soluzioni normative in termini di sospensione dei processi e di sospensione dei termini, soluzione alla quale abbiamo cooperato e che trova la nostra soddisfazione, salvo che su un punto marginale - che deve vedere il coinvolgimento di tutte le di tutte le componenti dell'amministrazione della giustizia. Non si ritiene congruente il riferimento a suggerire al Parlamento o al Governo? Togliamolo, ma che sia utile, direi necessario, accogliere questa istanza, che è pervenuta in più circostanze nelle assemblee che si sono tenute su questa materia, per fare in modo che vi sia un pieno coinvolgimento degli operatori della giustizia alla ripresa

Stiamo parlando di un'attività di sostegno al Governo, al Ministero, al consiglio giudiziario, al fine di risolvere i gravi problemi che ci sono.

Signora Presidente, volevo semplicemente osservare che sono le ore 20,10, quindi, se ella dovesse decidere comunque di andare avanti con l'illustrazione degli emendamenti, non credo che si potrebbe procedere al voto.

un problema che è stato evidenziato sul quotidiano «la Repubblica» questa mattina, con particolare risalto nelle pagine genovesi ma anche con un richiamo nelle pagine nazionali. pagine nazionali. Non ho motivo di pensare che le notizie riportate non siano corrette, anche perché ho avuto modo di parlare con alcuni insegnanti ed alcuni responsabili

tre istituti, che sono sotto un'unica presidenza - l'Istituto Einaudi, l'Istituto Casaregis e l'Istituto Galilei - la preside si è recata nelle classi in cui ci sono ragazzi stranieri,

Cosa sta succedendo? Mi dicono che ci sono situazioni in cui dei ragazzi che stanno per compiere 18 anni di età cominciano a non andare a scuola. scuola. Ho presentato un'interrogazione al ministro Gelmini perché ovviamente voglio capire se il fatto è veramente accaduto, se ci sono disposizioni ministeriali che inducono i presidi o gli insegnanti a individuare eventualmente

che possono trovarsi in questa condizione perché magari i genitori non hanno più il permesso di soggiorno o per tanti altri motivi e sappiamo che questo può essere anche un problema per affrontare la maturità.

che stanno per compiere 18 anni, di fronte alla possibilità di decidere di non andare più a scuola. E questo pensiamo possa servire all'integrazione o a dare maggiore sicurezza? Mi auguro che

in maniera incessante, pedante, ossessiva, probabilmente anche noiosa per alcuni, siamo intervenuti da questi banchi come delegazione radicale - in particolar modo lo ha fatto il senatore Perduca che oggi sostituisco indegnamente - per ricordare e denunciare come il Parlamento, le istituzioni debbano essere le prime a rispettare le leggi che si danno.

La conferma ci è arrivata dal sondaggio Crespi sulle elezioni europee che ribadisce ciò che andiamo sostenendo:

molti giorni - troppi - Marco Pannella è in sciopero della fame, ma da quattro è in sciopero totale anche della sete, per ricordare a noi, a se stesso e a chi

in Aula per l'approvazione del disegno di legge sull'energia nucleare, a convocare immediatamente un tavolo coinvolgendo i dirigenti della FIAT e i sindacati rappresentanti dei lavoratori,

giorni durante la manifestazione di Torino, a convocare le parti e a fare in modo che la FIAT parli, con chiarezza, rispetto al futuro di queste due grandi strutture, sia quella di Pomigliano d'Arco che quella di Termini Imerese.